nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

senatore Della Vedova, mi ritrovo nelle parole del collega Caliendo e del collega Casson. È una questione di *fair play*: ci si mette d'accordo, lo avevamo detto esplicitamente. Altrimenti,

Signor Presidente, anch'io voglio unirmi alle considerazioni dei colleghi. Quale Vice Presidente della Commissione ambiente vorrei giustificare i colleghi che non erano presenti perché impegnati in Commissione.

Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie ‑ PSI, voglio ringraziare in modo non formale la Commissione e la sua

Sarò breve, per non ripetere i punti già sollevati in discussione generale. Pongo tre piccole questioni. La prima: molti parlamentari che hanno un'esperienza molto maggiore della mia all'inizio di questo percorso di riforme, di fronte al mio entusiasmo, mi hanno sempre messo in guardia sul fatto che tanto sarà l'ennesimo tentativo destinato a finire nel nulla. Chi ne ha viste già tante prima può testimoniarlo.

appello, proprio perché non ci possiamo più permettere i costi economici, sociali e culturali, anche, di un sistema istituzionale inefficiente. È vero che viene sempre fuori qualcosa di più urgente all'ultimo minuto, ma questa volta francamente non dobbiamo permettere che accada. Il programma del lavoro del Comitato è molto ambizioso. È anche vero che più si mette carne al fuoco, più c'è il rischio che qualcosa vada vada storto e che fallisca. Mi riferisco soprattutto alla questione della legge elettorale, che, non a caso, ha occupato gran parte del tempo della discussione generale, anche se, in realtà, dal punto di vista istituzionale è un aspetto assolutamente minore. Il punto fondamentale mi pare sia la necessità di garantire la sistematicità del lavoro che il Comitato dovrà produrre, anche con riferimento al collegamento che questo avrà, naturalmente di tipo solo informale, con il lavoro del Comitato di esperti insediato al Governo. Per questo auspico che si arrivi non a quattro testi di revisione, magari coordinati nel modo più sistematico possibile, ma

è cambiato moltissimo da quando si è partiti, soltanto due mesi fa. Ieri il Ministro ci ricordava che l'ipotesi iniziale era quella di una Convenzione. Dico una cosa forse poco ortodossa in quest'Aula: personalmente ritengo che forse quella sarebbe stata l'idea migliore per garantire sistematicità (certo, avrebbe creato altri problemi sotto il profilo della legittimazione). Siamo arrivati al testo che abbiamo prodotto.

È giusto, però, vedere nel procedimento che si andrà ad approvare un atto di fiducia molto importante nel Parlamento, che il Parlamento, però, non potrà tradire. Come dicevo prima, questa volta non si può fallire. Si sono trovati degli equilibri molto difficili tra la centralità del Parlamento, da un lato, e la necessità di garantire quelle esigenze di pluralismo, di partecipazione popolare e di attenzione agli aspetti, anche tecnici e non soltanto politici, che sono necessari, Questi equilibri sono il frutto di un compromesso. Come tutti i compromessi, non c'è mai nulla di perfetto, ma il punto fondamentale su cui siamo chiamati a decidere in questo momento mi pare sia soltanto uno: Siamo d'accordo almeno sul fatto che la Costituzione richieda delle modifiche nell'interesse generale, generale, oppure no? Abbiamo almeno un minino comun denominatore, oppure no? Altrimenti è difficile anche partire. Occorre sfruttare l'occasione della grande coalizione che, in altri Paesi, di solito è la condizione ideale per produrre delle grandi riforme costituzionali: in Italia speriamo che lo sia. all'ultimo punto. Nel merito non entro, perché questa è una legge procedurale. Si tratta del metodo giusto per iniziare: iniziare dalla procedura e non dai contenuti. per il fatto che stiamo parlando di una legge procedurale - mi pare che i timori che sono stati avanzati in sede di discussione generale di un possibile eccesso del potere di revisione costituzionale siano, almeno in questa fase, del tutto infondati. Anche perché, come è stato richiamato anche dal senatore Campanella in sede di discussione generale, la Corte costituzionale ha affermato il proprio potere di sindacare la legittimità costituzionale di revisioni costituzionali qualora queste vadano ad infrangere La legge procedurale, però, non è soltanto tale, perché ci dà anche il perimetro del lavoro del Comitato, e ci sono alcuni aspetti che rischiano di minacciare un po' la sistematicità del lavoro. è la possibilità che si arrivi a quattro diversi testi che, magari soggetti a *referendum*, potrebbero portare a degli esiti diversi, con delle conseguenze sistematiche piuttosto disastrose. L'altro è - faccio soltanto

più garantito e per dire che è una deroga *una tantum* all'articolo 138. Tuttavia, da accademico dico che poi bisogna sempre cercare di trovare un senso alle parole del legislatore. In questo caso, il senso effettivamente è un po' pleonastico. comunque fondamentale partire e, poi, concentrarsi sui contenuti, sperando anche in modo costruttivo. Accenno soltanto alla questione della possibile - anzi certa - revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, relativamente ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali. Certamente noi ci batteremo affinché non prevalga quell'equivoco centralista che ogni tanto in questo Parlamento aleggia, secondo cui lo Stato potrebbe gestire meglio delle Regioni la complessità di cui si nutre questo Paese. Credo che questo sia un errore grossolano, e ci impegneremo affinché non trovi posto nei lavori del Comitato. In conclusione, mi pare l'elemento fondamentale sia soltanto uno: che ci voglia un minimo di condivisione nelle regole di fondo per fare una riforma costituzionale è una cosa ovvia, ma facciamo bene a ripetercelo. Non dobbiamo diventare - o sperare di diventare - improvvisamente come i britannici, che hanno una Costituzione talmente che non ha bisogno nemmeno di essere del tutto scritta, e quindi è rigidissima nella sua massima flessibilità. Noi, però, stiamo dando un po' prova di un eccesso di sospetto costituzionale, che produce anche un eccesso di regolamentazione. Concludo

e, in tal caso, un senatore e un deputato». È un dettaglio, un assoluto dettaglio, ma è rivelatore del fatto che non funzionano le convenzioni costituzionali, che non ci si fida di niente e di nessuno. Era chiaramente una norma implicita che si è voluto esplicitare proprio per questo eccesso di sospetto costituzionale. Ma allora è proprio per questo che la riforma è indispensabile, perché la nostra Costituzione, come sappiamo, soprattutto in tema di forma di Governo, è a maglie molto larghe e presuppone molte convenzioni. Se non siamo in grado di riempire queste maglie con un comportamento di fiducia reciproca, a maggior ragione abbiamo bisogno di una Costituzione che sia più puntuale e più dettagliata e che possa prevenire

*(GAL)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe, colleghi, siamo arrivati nei tempi sufficientemente celeri che ci eravamo prefissati a questo primo appuntamento: si dà avvio dà avvio al progetto di revisione costituzionale e si organizzano i primi strumenti per poter rendere efficace, importante, la riforma che ci accingiamo Non potremmo che essere che soddisfatti, anche se la soddisfazione deve lasciare posto anche ad alcune puntualizzazioni che si rendono necessarie per il prosieguo della nostra azione. In questi giorni esercitare vizi privati e pubbliche virtù. Abbiamo assistito ad una Commissione che ha molto lavorato e che al suo interno ha trovato delle mediazioni importanti. Noi stessi, Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, abbiamo presentato l'emendamento 2.22 che

Con questo stesso spirito di fattività e collaborazione hanno lavorato tutti gli altri Gruppi, anche coloro che si sono dichiarati contrari a questo processo di revisione costituzionale, tranne poi registrare comportamenti in Aula o sulla stampa diversi da quelli che abbiamo potuto constatare nei tavoli di lavoro. Ho potuto assistere a un intervento piuttosto appassionato, ma devo dire un po' ipocrita, dal mio punto di vista, di un rappresentante del Gruppo Misto, che è arrivato a dire che avremmo dovuto occupare meglio il tempo a nostra disposizione per risolvere i problemi economici del Paese, dell'occupazione o della disoccupazione, quasi che chi si voglia porre il problema della riforma costituzionale non abbia a cuore questo tipo di questioni. Ma quante volte ce lo siamo detto, senatore Uras, che anche la riforma costituzionale è un momento importante, fondamentale, dello sviluppo economico, quello e dello svecchiamento delle nostre istituzioni? Quante volte ce lo siamo detto? di dieci minuti di intervento in Aula, che pensiamo possa captare la benevolenza di chi ci ascolta, riusciamo a demolire anche quello che riusciamo a fare in Commissione in uno spirito

e una gestione più moderna della nostra Nazione e della nostra Italia, sono qui a tenere atteggiamenti un po' ostruzionistici e ad inserire elementi...

delle dichiarazioni pubbliche e dei comportamenti che si realizzano di conseguenza? Ieri abbiamo ascoltato il capo del Movimento 5 Stelle Grillo

gli atteggiamenti tenuti in Aula, ad esempio, dal senatore Crimi, in merito alla questione della giustizia: ieri ha addirittura invocato allo scandalo, allo scalpore, perché in quest'Aula si ponevano i problemi della giustizia del singolo o di quell'altro. Mettiamoci d'accordo su un fatto, cari amici. Indigniamoci per le cose che davvero ci fanno indignare moralmente e dall'interno. Quando si affrontano le riforme, quando si vuole fare un servizio al Paese, Paese, lo si rende in maniera piena, se riusciamo a discernere la propaganda, il momento di proselitismo o di campagna elettorale da quello che è sostanza, da quello che è necessario. Anche sul necessario ci si può dividere, perché le ricette per il meglio possono

Lo abbiamo già lamentato all'inizio del percorso. Non abbiamo avuto il coraggio di affrontare il problema del Titolo IV della Costituzione, il problema della giustizia. Lo abbiamo escluso dal novero dell'azione

del sistema della giustizia nel nostro Paese. Porremo attenzione a tutto questo. Intanto si parte. È importante partire in tempo. È importante partire con coesione.

di taluni aspetti ma il processo costituente non può che coinvolgere tutti quanti. Anche il Governo, onorevole Ministro, deve essere più attento.

Non ci è piaciuto, anche perché talvolta la fretta è cattiva consigliera. Anche nella stessa formulazione si sarebbe dovuti essere più attenti, signor Ministro, perché lei... Ministro, il collega Mauro richiede la sua attenzione, giustamente. La ringrazio, signor Ministro. M5S).* La crassa risata del collega pentastellato è proprio un piacere, ridondante nella nostra Aula. Come dicevo, signor Presidente, gli effetti annuncio non servono, neanche quando provengono dal Governo, perché abbiamo bisogno di riforme armoniche.

annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, augurandoci che questo grande progetto di riforma costituzionale potrà portare al rinnovamento del nostro Paese.

e durante la votazione degli emendamenti abbiamo avuto modo di porre una serie di questioni per noi assolutamente fondamentali, e quindi di sottolineare ampiamente i punti che, a nostro avviso,

elemento forte e importante anche per il futuro del nostro Paese. Anche allora si definirono innovatori i componenti di quella maggioranza, che votò

Non ci sentiamo neanche conservatori - lo dico con molta franchezza

per modificare la Costituzione in alcune parti in modo puntuale, preciso e circoscritto (ma

alla costituzione del Comitato - quali sono effettivamente le questioni che si ritengono più urgenti, qual è il limite cui si vuole arrivare e dove ci si vuole spingere.

purtroppo, questo dibattito un po' frettoloso - ne hanno parlato anche altri senatori - non è una novità nel nostro Paese. Il senatore Tocci l'altro giorno parlava di una sorta di ossessione compulsiva alle riforme. Condividiamo in pieno, anche perché non ci sembra che questa ossessione compulsiva abbia prodotto ad oggi

la responsabilità del malfunzionamento della nostra democrazia, del distacco enorme tra i cittadini, la politica e le istituzioni: responsabilità che è invece tutta quanta in capo alla malapolitica. E non sto parlando genericamente di autoriforma, ma la dico così com'è: la cattiva politica.

come se quello che è accaduto in quei giorni fosse responsabilità della Costituzione. Invece, come sappiamo perfettamente, era responsabilità della cattiva politica, e non voglio aggiungere altro. altro. È questo autoassolversi, cercando di buttarla sulla Costituzione e sulle riforme, magari come panacea di tutti i mali, che non condividiamo affatto.

alla centralità del Parlamento. Abbiamo discusso questa mattina in modo ossessivo, e non avete voluto modificare questo punto assolutamente fondamentale sul diritto di ogni parlamentare di poter partecipare al procedimento e quindi di poter presentare subemendamenti, e non è una questione secondaria.

solo ed esclusivamente della maggioranza. Ma non vi porterà bene: ricordate la fine che hanno fatto gli altri tentativi di riforma da questo punto di vista. La verità - e termino il mio intervento, Presidente, dichiarando il voto contrario delle senatrici e dei senatori del Gruppo Misto Sinistra Ecologia

nel giorno dell'insediamento del vostro Governo, la Lega Nord ha espresso un voto di astensione perché il presidente Letta, nel suo intervento, ha saggiamente parlato di riforme e di tempi certi per la loro realizzazione. Ora però, dopo tre mesi, è giunto il momento di fare un bilancio, sia rispetto all'azione generale di governo, sia rispetto al fronte delle riforme. Caro ministro Quagliariello, il Governo a cui lei appartiene e la maggioranza che lo sostiene sono un vero disastro. Non ho mai visto una maggioranza così ampia di Governo e così sgangherata, ma non ho neanche mai visto che a sparare ogni giorno addosso al Presidente del Consiglio o ad uno dei suoi Ministri siano i più alti esponenti dei partiti che compongono la compagine di Governo.

non sembrano esserci solo i partiti di maggioranza, sembrano esservi anche alcuni Ministri e Sottosegretari che, parlando a vanvera e a ruota libera, dimostrano la loro inadeguatezza rispetto al ruolo che ricoprono e mettono oggettivamente in difficoltà il Presidente del Consiglio. Ma lasciamo perdere le persone e andiamo ai contenuti. I provvedimenti assunti sull'IMU e sull'IVA sono una vera barzelletta. Piuttosto che abolire definitivamente l'IMU, come noi avevamo fatto con l'ICI, e cancellare l'incremento dell'IVA, le avete solo rinviate, e tra l'altro l'avete fatto senza copertura. Uno Stato che per rinviare l'incremento di un'imposta chiede l'anticipo di un'altra imposta, pari o superiore al cento per cento, sta facendo una rapina di Stato nei confronti del cittadino. *(Applausi

l'azione di governo è una tragedia: il vostro motto è non decidere, differire, spostare, non fare. «Sopire, troncare, (...) troncare, sopire» avrebbe detto il vecchio conte zio de «I Promessi Sposi».

lo avete dimostrato quando bisognava fare le nomine: su quelle al primo colpo avete trovato la quadra e avete sistemato tutti nel cimitero degli elefanti della pubblica amministrazione, amici e parenti, con buona pace dei debiti pubblici e della meritocrazia. Lo stesso decisionismo l'avete dimostrato solo quando avete fatto un decreto-legge per far uscire dalle carceri migliaia di delinquenti *(Applausi dal di tornare a delinquere, visto che si tratta anche di recidivi. Caro Governo, il numero e la capienza delle carceri vanno parametrati al numero dei reati commessi e non il contrario. Se una buona parte della popolazione carceraria è costituita da cittadini extracomunitari o stranieri, che vadano a scontare la pena nel Paese di provenienza risolvendo da una parte il problema del sovraffollamento carcerario e, dall'altra, liberando risorse che rendano la detenzione uno strumento di rieducazione e riabilitazione e non solo di punizione. Ma lasciamo perdere l'azione generale di governo (ci vorrebbero dei giorni per commentarla). Purtroppo, anche sulle riforme rischiamo di andare per le lunghe. Letta nel suo discorso aveva parlato di diciotto mesi per realizzarle, ma da allora sono già trascorsi tre mesi, e siamo già a ventuno mesi, ai quali bisogna aggiungere i quattro mesi necessari all'approvazione del Comitato, e siamo così arrivati a superando in questo modo anche il periodo di gestazione di un pachiderma. Di più, il testo originario del Governo parlava di «assicurare» entro diciotto mesi il varo della riforma, mentre il testo della Commissione è passato ad un più debole «consentire», che in termini di certezza dei tempi - mi consenta - mi fa venire in mente la battuta «mia figlia è incinta, ma solo un pochettino». io continuo a crederci, nonostante solerti convocazioni di altre Aule sembrino dimostrare il contrario. Caro senatore Mauro, non è vero che non si è parlato di Titolo IV della Parte II della Costituzione: ieri abbiamo occupato la giornata a parlare del Titolo IV. Noi abbiamo dato un contributo in Commissione facendo approvare numerosi nostri emendamenti che hanno reso certi il Comitato e la sua operatività, e il nostro contributo abbiamo continuato a darlo anche in quest'Aula con tanti ordini del giorno che pongono paletti per la prossima scrittura della riforma. Ma quando arriveremo al dunque non dovrete, né potrete, tradire la nostra fiducia. Cara presidente Finocchiaro, caro ministro Quagliariello, fatevi tanti bei nodi al fazzoletto quanti sono i punti che ora andrò ad enunciarvi. Primo: il numero dei parlamentari non va ridotto per finta, va dimezzato veramente, tenetelo a mente. fra deputati e senatori bastano e avanzano. Secondo: il Senato federale. Il presidente Letta nel suo intervento ha parlato di un vero Senato federale, come noi lo vogliamo, e non di un papocchio fatto solo per accontentare gli attuali senatori o chi lavora nel Palazzo. Terzo: premierato forte o semipresidenzialismo. Personalmente non sono innamorato di uno dei due modelli, ma pretendo una formula che preveda che il Governo possa governare, che il Parlamento possa legiferare e indirizzare l'Esecutivo e che l'opposizione possa svolgere la propria funzione di controllo e di garanzia. Quarto: federalismo. Ma questa volta lo si faccia veramente stabilendo, una volta per tutte, che cosa deve fare lo Stato, che cosa devono fare le Regioni e che cosa gli enti locali. Ma attenzione! Non vorrei mai che qualcuno tentasse, con la scusa di mettere ordine al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, di riportare tutto in capo allo Stato cancellando quel po' di federalismo presente nella nostra Costituzione.

Le bozze che escono clandestinamente dal suo Dipartimento non ci piacciono, glielo dico chiaro: Ministro avvisato, Ministro mezzo salvato. federalismo fiscale. Questa riforma dovrà, come ha detto il presidente Letta, stabilire una più equa ripartizione delle entrate fiscali fra centro e periferia, e dovrà essere l'occasione per dare piena attuazione al federalismo fiscale approvato nella precedente legislatura, a partire dai costi *standard* incredibilmente messi nel cassetto dal Governo Monti. Se venissero applicati anche solo i costi sanitari *pro capite* della Regione Lombardia in tutte le Regioni, avremmo un risparmio strutturale di 27 miliardi di euro all'anno: Sesto: a noi interessano anche le macroregioni, che non dovrebbero interessare solo al Nord ma anche e soprattutto al Sud e a quelle Regioni

Basta con la politica degli annunci e testi scritti in fretta, che fra l'altro, con le norme transitorie, rimettono in essere come prima le vecchie Province! Si legga piuttosto la mia proposta, che le trasforma in enti locali regionali, la cui competenza ordinamentale esclusiva spetterà alle Regioni. Ciascuna Regione dovrà e potrà decidere sul numero e sul ruolo delle Province in base alle proprie necessità: questo è federalismo!*(Applausi noi voteremo sì a questa legge, ma da ora partirà il *timer*, che per lei e per il presidente Letta sarà il *timer* di una bomba a mano: se non si dovessero realizzare le riforme nei termini stabiliti

per il lavoro che hanno svolto e per la sensibilità con la quale hanno affrontato questo argomento così importante per tutti noi. Quella di oggi potrebbe essere un'occasione formale: poter dire di sì a un disegno di legge che è meramente procedurale. Ma sappiamo che non è così, iniziamo un cammino difficile e probabilmente avrà ragione lei, senatrice De Petris, a dire che questo percorso riformatore è solo una polizza sulla vita del Governo. Purtroppo altre nubi si addensano all'orizzonte, e ci auguriamo che il comune riferimento ai valori fondanti della Repubblica, tra cui il principio della separazione dei poteri, aiuti a non offuscare la saggezza e la prudenza dimostrate sin qui da chi pure si richiama alla tradizione liberale e ha in questa tradizione i propri riferimenti ideali. Ma ben venga questa polizza sulla vita, se è tale da darci tra poco più di un anno un Parlamento profondamente rivisitato, ridotto nelle sue dimensioni ma potenziato nell'efficienza e nell'efficacia, saldo nella sua centralità rispetto alle altre istituzioni. Ben venga, se è tale da darci una Costituzione che riscriva il rapporto tra Stato centrale e autonomie, superando la schizofrenia di questi dieci anni portata avanti spesso violentandola proprio in nome delle autonomie. Ben venga se, con un Governo che recupera piena legittimazione democratica e con una legge elettorale più rispettosa dei diritti degli elettori, la politica riuscirà a ricucire un rapporto fiduciario, oggi lacerato, con il Paese. Rattrista, quindi, sentire soprattutto da chi non perde occasione per ricordare la centralità del Parlamento commenti, critiche, attacchi, parole, a volte anche fuori di senno, contro quello che stiamo facendo in questi giorni. Stiamo facendo esattamente quello che abbiamo promesso durante la campagna elettorale per recuperare una credibilità compromessa: avviare, cioè, una riforma costituzionale per dare all'Italia istituzioni più efficienti ed efficaci, ma altrettanto rappresentative, e per consentirci di mantenere il posto che ci compete in Europa e nel mondo. Certo, siamo solo all'inizio. Il percorso non sarà breve; molto e molti cercheranno di interromperlo o di ostacolarlo. Siamo però consapevoli che sul raggiungimento di quest'obiettivo non solo la maggioranza, ma tutto il Parlamento misurerà la propria credibilità. Non possiamo permetterci di fallire. Incombe sulla maggioranza il dovere di fare in modo che questa priorità, indicata dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio in occasione della loro investitura, non venga disattesa. Con il voto a favore di questo disegno di legge, Scelta Civica per l'Italia intende aderire senza riserve a questo che per noi è un dovere non solo di lealtà verso il monito della più alta magistratura della Repubblica o verso un Governo, ma di coerente fedeltà a un patto che abbiamo scritto il 25 febbraio con tre milioni e mezzo di elettori. *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, signori del Governo, siamo arrivati quasi alla fine della procedura d'urgenza con cui quest'Aula ha deciso di trattare il disegno di legge per l'istituzione del Comitato per le riforme costituzionali. Il Movimento 5 Stelle crede che la Costituzione vada aggiornata per ottimizzare gli organi e le procedure che vi sono previsti, per renderli più efficaci e per ridurre i costi della macchina dello Stato. Ma non è solo una considerazione di ordine economico, piuttosto un'esigenza sociopolitica: evitare la costituzione ed il mantenimento di un ceto che gestisca la cosa pubblica e tenda a costituirsi come un corpo separato, come una vera classe. Invece i partiti, che negli ultimi venti-trent'anni non sono riusciti a gestire l'ordinario, si ripromettono e promettono al popolo italiano di fare cose straordinarie. Il Movimento 5 Stelle crede che nell'ordinamento disegnato dalla Costituzione debbano essere iniettate robuste dosi di democrazia diretta e di ogni accorgimento idoneo a restituire realmente il controllo dei processi politici ai cittadini. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle è contrario alla costituzione di questo Comitato. Le ragioni le abbiamo analizzate nelle ultime settimane nei nostri interventi in Commissione e in Aula. Permettetemi ora di sintetizzarle. Uno dei problemi è l'origine politica di tale Comitato, che è molto, molto legata alla composizione politica della strana maggioranza che regge l'attuale Governo. Tale maggioranza ha voluto raccogliere l'invito del Presidente della Repubblica a realizzare le riforme, ma forse non ha colto un aspetto nodale. Il risultato elettorale, che è alla base della composizione di questo Parlamento, è stato un campanello d'allarme fortissimo per i partiti politici che da decenni occupano e gestiscono le istituzioni. La risposta è stata la dichiarazione di volontà di realizzare le riforme. Attenzione: è una dichiarazione di volontà, ma di sola volontà, o sola dichiarazione, perché non c'è un'intesa di massima tra le forze presenti in Parlamento, ma non c'è un'intesa di massima neanche tra le forze presenti nella maggioranza. Noi sappiamo che una parte non ha alcuna intenzione di accedere a forme presidenzialistiche o semipresidenzialistiche e un'altra parte è proprio quelle che vuole.

dove il Titolo IV, per i cittadini che ci ascoltano, è la magistratura. C'è una parte di questo Parlamento che, nella maniera più trasparente e chiara possibile, ha manifestato l'intenzione

è liberale in modo flessibile. È liberale per la parte che le interessa, lo è meno quando si parla di divisione dei poteri. A questo punto, l'intesa tacita sembra essere quella di prendere tempo, prendere tempo, per dare luogo all'attività di un Governo in un momento di obiettiva difficoltà economica, fortissima per l'Italia ed estremamente sentita tra i cittadini, tra i cittadini, per non affrontare il tragico nodo della riforma elettorale, che è un altro dei pomi della discordia, perché siamo stati abituati da anni a vedere riforme elettorali che servivano gli interessi della parte che se ne faceva promotrice. questo punto, quindi, noi prendiamo la riforma elettorale da farsi (perché che si debba fare è chiaro a tutti, soprattutto ai cittadini), e la spostiamo a data da definirsi,

la volontà di rispondere alle esigenze dei cittadini. Signori, noi sappiamo tutti qua dentro, come lo sanno fuori, che i cittadini questa drammatica esigenza

come poc'anzi ricordavano i colleghi della Lega: il numero dei parlamentari. E anche quella è un'esigenza legata non ad una consapevolezza dell'eccesso del numero, quanto alla quanto alla consapevolezza dell'improduttività delle Aule parlamentari negli ultimi anni. Il problema però non è che le Aule parlamentari sono improduttive perché piene di membri che non sono capaci di operare: le Aule parlamentari sono improduttive per motivi che sono stati chiarissimamente esemplificati ieri pomeriggio. Sono improduttive perché da una parte c'è l'interesse, oramai conclamato, reso assolutamente patente, a difendere una persona: non un principio, attenzione, perché ai difetti del malfunzionamento della giustizia ci sono moltissime persone in Italia che sono assoggettate, sia che si tratti di giustizia penale, sia che si tratti di giustizia civile. Però alla giustizia, anche a quella minima del giudice di pace, normalmente si risponde mettendo un balzello per accedere alla pronuncia del giudice di pace. quindi, un'esigenza avvertita allo stesso modo da tutti. Quindi, colleghi del PdL, quando dite che si tratta di assicurare giustizia a ciascun cittadino, non è così, perché parliamo di un cittadino chiarissimamente e personalmente definito, che conosceremmo tutti meglio se fosse più presente in quest'Aula. A questo punto, in questo stato di cose, la prima vittima è la rigidità della nostra Costituzione, rigidità che i Padri costituenti avevano posto a guardia del funzionamento della Repubblica, che deve essere fondato su alcuni punti fermi. fermi. Il bello, la caratteristica della Costituzione è che ci dà una griglia all'interno della quale poterci muovere anche con la normazione. Noi, invece, questa rigidità, nel momento in cui più serve e nel momento in cui meglio deve essere affermata, affermata, la mettiamo da parte per far prima e per far meglio. Come? Riducendo le prerogative dei parlamentari; riducendo i tempi tra una lettura e l'altra delle leggi costituzionali che eventualmente si approvassero; sostanzialmente comprimendo la funzione del Parlamento, anche a vantaggio del Governo che improprissimamente - mi si perdoni il termine - viene chiamato ad agire nel processo proponendo un disegno di legge e chiamando a raccolta un gran numero di accademici per consigliarlo...

è stato detto in maniera chiara, netta, limpida che c'è un problema nella composizione di questo Parlamento. Non si tratta di un problema formale, ma sostanziale, nella misura in cui nessuno di noi presenti in quest'Aula è stato direttamente votato da un cittadino.

e concludo, signor Presidente. Abbiamo provato a contribuire chiedendo una maggiore partecipazione ai cittadini e continueremo a farlo. Quest'Aula si è impegnata con l'approvazione di un ordine del giorno. Cercheremo di realizzare effettivamente questa cosa. Quest'Aula, ripeto, si è impegnata e a questo punto noi speriamo di ridurre il danno, perché siamo consapevoli che all'interno di quest'Aula siamo in netta minoranza, ma siate consapevoli che che all'esterno di quest'Aula siamo altrettanto nettamente maggioranza. *(PdL)*. Signor Presidente, mi preme da subito affermare che noi voteremo a favore di questo provvedimento. La prima motivazione che ci vede favorevoli è quella che inerisce e riporta, con questo provvedimento, la centralità del Parlamento. Ricordo quando, all'inizio di questo dibattito, taluni avrebbero voluto un Comitato composto da membri del Parlamento e da membri cosiddetti laici. Non se ne comprendeva a fondo l'intenzione dei proponenti, ma fortunatamente tale percorso è stato accantonato. Mi sia consentito aggiungere sul punto un'ulteriore considerazione. Non comprendo a quale fine il Governo ha invece optato per la costituzione nel suo seno di un collegio dei saggi, che dovrebbe avere la finalità di collaborare per la migliore redazione dei testi che il Governo poi offrirà al Parlamento stesso. L'esperienza maturata già alla Camera dei deputati, ma anche quello che è avvenuto nella Commissione affari costituzionali del Senato in sede di audizione

due professori universitari, che mi sento di ringraziare per il loro rigore scientifico e per la loro profondità; ma sia il professor Pace che il professor Marini ci hanno illustrato tesi contrastanti che, se amplificate in un consesso di 42 esperti, poco o nulla potranno concorrere per facilitare e supportare l'attività del Governo e conseguentemente l'attività del Parlamento. D'altra parte i *rumors* di queste ore circa le differenti posizioni di questi saggi confermano l'assunto superiore. Ma tant'è: quella scelta il Governo l'ha fatta e attendiamo fiduciosi, anche se con una punta di scetticismo, il lavoro che si sta producendo. Tornando al nostro disegno di legge, sottolineo che trattasi di un provvedimento che si prefigge di fissare le linee guida, le regole, l'*iter* che dovrà essere osservato per pervenire alle auspicate riforme della Parte II della Costituzione. Il testo offertoci dal Governo era già in linea di massima condiviso e si è cercato di lasciarlo, il più possibile, com'era nella sua stesura originaria, salvo intervenire su determinati punti, solo per renderlo più rispondente al dibattito che si è sviluppato in Commissione, sia in sede di discussione generale sia in quello che è scaturito nella fase emendativa. In particolare, abbiamo ritenuto, come PdL, di presentare pochi emendamenti che completassero e meglio definissero taluni passaggi che il Governo aveva ipotizzato. Concretamente, abbiamo ritenuto che non fosse abbastanza chiara la lettura del testo nella parte che indicava la composizione numerica del Comitato. Un nostro emendamento ha meglio specificato che ai quaranta componenti dovevano aggiungersi i due Presidenti delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Poi abbiamo ritenuto che, in assenza di riferimenti alle modifiche necessarie al Titolo IV e VI della Parte II della Costituzione, si poteva concretizzare il dubbio che comunque il Comitato non sarebbe potuto intervenire su quelle parti, appunto del Titolo IV e VI, per le correzioni che si fossero rese necessarie a seguito delle modifiche sulla forma di Stato e sulla forma di Governo. Basti pensare alla Presidenza del CSM oppure al criterio di nomina dei giudici della Consulta, laddove dovessimo decidere sulla fine del bicameralismo perfetto, che vedrebbe quasi certamente il Senato titolare di un proprio diritto circa la nomina di un numero da stabilirsi dei componenti della Corte costituzionale. Altro punto da noi ritenuto qualificante è stato quello relativo all'esame dei progetti di legge aventi ad oggetto la riforma della legge elettorale che necessariamente dovrà essere conseguente al nuovo assetto che nel merito il Parlamento andrà a decidere. E ciò fermo restando che alle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato non è preclusa la possibilità di discutere e valutare leggi elettorali che venissero ritenute necessarie e opportune, valutazione, peraltro, tutta politica. Sconsiglierei, sul punto, fughe in avanti, se non concordate in sede politica, perché queste potrebbero avere il solo fine di far collassare il processo riformatore. Altro punto di particolare importanza è rappresentato dall'articolo 5, che attiene al *referendum*. Si è voluto rafforzare la portata dell'articolo 138 della Costituzione, prevedendo, se richiesto, il *referendum* anche quando la legge è stata approvata con il *quorum* dei due terzi. In conclusione, sento di dover ringraziare tutti coloro che sono intervenuti sia in questa sede, sia in Commissione. In particolare, un ringraziamento mi sia consentito alla relatrice presidente Finocchiaro e al ministro Quagliariello. Ho ascoltato tanti interventi che ci hanno intrattenuto anche toccando questioni di merito, in questa sede certamente fuori luogo e ultronei: ci sarà tempo e tutti gli argomenti che dovranno essere trattati saranno sviluppati degnamente. Insisto: questo è un provvedimento teso solo ed esclusivamente a stabilire regole e procedure da porre a base del gravoso lavoro che ci attende. Quello odierno è il secondo gradino, dopo l'approvazione della mozione sulle riforme costituzionali del 29 maggio 2013, a cui seguirà quello dei testi sulla nuova configurazione dell'assetto istituzionale. Mi auguro che il processo riformatore questa volta possa procedere senza intoppi per giungere a conclusione. Sarebbe la scrittura di un bel libro: oggi stiamo tutti insieme scrivendo una pagina importante ed io - personalmente - ne sento anche la responsabilità.

ma non sono nemmeno delle modifiche sostanziali della nostra Costituzione, come dicono altri. Politicamente, nella sostanza, esse segnano l'avvio di un percorso di riforma i cui contenuti debbono essere ancora elaborati e definiti. Nel metodo, vedo nel provvedimento rilevanti indicazioni di fondo: la conferma della necessità di rispettare lo spirito e le prescrizioni dell'articolo 138 ma anche la necessità e l'urgenza del processo riformatore. La decisione della Corte costituzionale sull'incostituzionalità della legge ordinaria di riduzione delle Province ci dice quanto poco servano le scorciatoie. Larga parte dell'opinione pubblica si chiede se il Parlamento sarà all'altezza di questo impegno, se saprà portare a compimento il processo riformatore. Non è una domanda ingiustificata, considerato quanto la politica del rinvio ha danneggiato l'Italia. Non parlo di rinvii di settimane o di mesi: parlo dei ritardi di decenni delle politiche di riduzione del debito pubblico, della soluzione del dramma dell'evasione e dell'elusione fiscale, della difesa dei beni culturali e del paesaggio, del rinnovamento della scuola pubblica, dell'ammodernamento dei servizi pubblici. signor Presidente, parlo dei ritardi della riforma della pubblica amministrazione, di azioni di contrasto alle oligarchie, di regolamentazione seria del conflitto di interessi. Da anni - ancora - rinviamo decisioni largamente condivise su limitate modifiche della Costituzione, come la riduzione del numero dei parlamentari,

Cosa è cambiato per poter dire che la politica del rinvio non sarà più la nostra? Ecco che cosa è cambiato: mentre noi restavamo fermi e ripiegati su noi stessi, è cambiato il mondo, e chi non lo comprende è destinato a soccombere. Oggi la violenza e la durata della crisi, la velocità dei fenomeni e una globalizzazione senza regole ci dicono che, se non saremo capaci di trovare in noi stessi, con i tempi rapidi dei mutamenti globali, la forza e le idee necessarie per battere le nostre malattie e i nostri vizi, saremo destinati inesorabilmente a perdere sovranità e a a ridurre il tenore di vita e i livelli di sicurezza sociale. In una parola, saremo destinati ad un declino rapido, violento e pericoloso. Lo dico al mio amico senatore Tocci: la difesa della democrazia da parte del Partito Democratico è fuori discussione. Ma lo è altrettanto l'urgenza di trovare soluzioni giuste ed efficaci ai nostri gravissimi problemi. io condivido l'analisi della presidente Finocchiaro: sarebbe molto, molto rischioso se nel Paese diventasse senso comune l'idea che il Parlamento è inutile. E lo dico anche, con molto rispetto, al Movimento 5 Stelle: io non mi scandalizzo per le proteste d'Aula; mi preoccupa la sensazione che pregiudizialmente

Ci sono aspetti della nuova normativa costituzionale, che tra poco approveremo in prima lettura, che hanno un rilevante significato politico. Il Comitato di deputati e senatori, cui pariteticamente è demandata l'elaborazione in sede redigente delle modifiche alla Costituzione, esprime, proprio per la sua composizione mista, una esplicita presa d'atto dei limiti del bicameralismo paritario disegnato nel 1947 dai Padri costituenti. E su questo punto serve una riflessione: non sul bicameralismo che nel 1947 venne scelto con molta saggezza, quanto sulla sua attualità oggi, dopo quasi settant'anni, in una fase storica molto diversa politicamente, economicamente e socialmente. Ma qui entriamo nel campo dei contenuti, sui quali dobbiamo aspettare le risposte del Comitato, a cominciare - lo ripeto ancora - da quelle sulle funzioni di Camera e Senato, sul numero dei parlamentari e sul Titolo V. Il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali prevede una specialissima composizione del Comitato: i suoi componenti saranno individuati secondo il duplice criterio della consistenza dei Gruppi e del numero dei voti conseguiti dalle liste. Mai, prima d'ora, era accaduto che una Commissione parlamentare non venisse composta, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, secondo la proporzione dei Gruppi parlamentari. Il Partito Democratico ha dato il suo consenso a questa modifica, così rinunciando al suo legittimo diritto di vedersi rappresentato in relazione alla sua forza parlamentare. Non ricordo casi nei quali altri Gruppi si siano comportati nello stesso modo. Ma tutti i senatori, non solo del Partito Democratico, hanno piena consapevolezza delle gravi ragioni che in queste circostanze impongono di violare, in via eccezionale, la necessaria proporzionalità che in Parlamento regola la composizione delle Commissioni; e la ragione sta tutta nelle gravissime conseguenze distorsive che il "porcellum" sta producendo alla nostra democrazia e che il Partito Democratico non vuole abbiano effetti sul processo di revisione della Costituzione. Presidente, le leggi elettorali sono formalmente leggi ordinarie, ma nella sostanza hanno indiscutibile valore costituzionale. Una buona Costituzione (e la nostra lo è) può perdere gran parte della sua forza democratica per una legge elettorale malfatta, fuori dai principi di una democrazia compiuta. Ed è per questo motivo, nel momento in cui si apre in Parlamento un dibattito sulla modifica di alcune parti limitate della Costituzione, che a nome dei senatori del Partito Democratico mi rivolgo all'intero Senato chiedendo che contestualmente venga data una priorità assoluta all'urgente modifica della legge elettorale vigente *(Applausi che ha già avuto effetti rovinosi e che non possiamo rischiare d'essere costretti ad utilizzare ancora una volta. Conosco l'obiezione che le leggi elettorali seguono e non precedono le riforme sull'assetto dello Stato e del Parlamento. È un principio talmente sacrosanto da farci dire che l'Italia avrebbe tratto grande giovamento se oggi chi di questo principio si fa scudo ne avesse tenuto conto anche nel 2005, quando il "porcellum" fu adottato a maggioranza, per freddo calcolo politico, senza che fosse intervenuta alcuna modifica dell'assetto istituzionale. Siamo in una situazione di grande pericolo. Sono gli italiani che ci chiedono all'unanimità di abrogare immediatamente il "porcellum", palesemente incostituzionale nel potere di scelta sottratto agli elettori, nell'abnorme premio attribuito senza condizioni, nei diversi sistemi tra Camera e Senato che determinano diverse maggioranze. Siamo in grave ritardo. Signori senatori, non usiamo strumentalmente l'alibi dei tempi lunghi del processo riformatore per condannare l'Italia all'umiliazione della peggiore legge elettorale d'Europa, totalmente estranea alla cultura giuridica e democratica della nostra Repubblica. Il Presidente della Repubblica, pochi giorni fa, ha sottolineato, con ragione, la necessità che il nostro Paese riacquisti fiducia in se stesso. La diffusa mancanza di fiducia, a cominciare da quella degli italiani nei confronti della politica, è uno degli elementi che più ci indebolisce di fronte alle difficoltà: sfiducia dei cittadini nelle proprie capacità ma anche, e assai prima, sfiducia nella politica e sfiducia nel Parlamento. Diciamocelo con chiarezza. Finché il Parlamento non si farà carico concretamente e sul serio dell'unanime richiesta degli italiani di abrogare il "porcellum", noi senatori e i nostri colleghi deputati non avremo alcuna possibilità di aspettarci la loro fiducia. Il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del provvedimento.

È una definizione semplificata, ma mi serve a far capire quella che per me è l'ipocrisia che sta alla base di questo ennesimo tentativo di modernizzare la nostra Carta costituzionale e che rischia di diventare il peccato originale, la lacuna che può determinarne l'inutilità. Perché parlo di ipocrisia? Perché, mentre noi qui parliamo di regole, la magistratura, o meglio una parte di essa, tenta di ridisegnare il sistema politico italiano, eliminando una delle rappresentanze popolari con una serie di inchieste e di processi in cui le regole vengono piegate a questo fine. Ma questa è solo una delle contraddizioni - per usare un eufemismo - del nostro sistema giudiziario. Le cronache, anche le più recenti, sono ricche di esempi: la vicenda controversa dell'Ilva ha messo in crisi una città; la condanna dei sismologi che non hanno previsto il terremoto dell'Aquila ha messo in crisi la Protezione civile; a Milano - notizia di oggi - uno stupratore non è andato in carcere perché una giudice, ad un anno dalla sentenza, non ne aveva ancora scritto le motivazioni. Ed ancora, una delle ragioni per cui grandi gruppi stranieri non investono in Italia è perché manca la certezza del diritto: un reato che non è non perseguito a Roma viene perseguito a Milano; un reato che è perseguito a Napoli non lo è a Siena. Più che un sistema giudiziario è una lotteria. Insomma, la nostra giustizia è malata. Qualcuno può anche non condividere questa lettura dei fatti, contestarla, dire che non è obiettiva o addirittura denunciare che sia una mistificazione. Quello che non si può fare, e che non può certo fare una classe dirigente, è accettare un compromesso al ribasso, o per ignavia o per assenza di coraggio. Decidere, cioè, che quell'argomento, ovvero i limiti e le distorsioni che riguardano il potere giudiziario, non debba essere toccato e non riguardi il legislatore, malgrado ne sia condizionato quotidianamente. Basta leggere l'editoriale di domenica scorsa di Galli della Loggia sul «Corriere della Sera» - buon ultimo, visto che non sono pochi quelli che lo dicono da anni - per scoprire che quella che stiamo mettendo insieme è una incongruenza. Galli della Loggia scopre per alcuni versi l'uovo di Colombo, ossia che nel nostro Paese Governo e Parlamento hanno solo il potere di proporre, ma che *lobbies*, burocrazia e potere giudiziario possono esercitare un potere di veto sulle loro decisioni e condannare il Paese all'immobilismo. Ebbene, decidendo di non affrontare la questione giudiziaria nella riforma costituzionale, di non aggiornare regole che ormai sono scritte solo sulla carta, ma che sono state reinterpretate nella prassi,

una sorta di casta, appunto - la vera casta - su cui non si può legiferare in Parlamento, ma solo magari attraverso *referendum*, il che, nei fatti, è il segno di un'impotenza istituzionale. quindi cambiando la forma di Stato e di Governo all'insegna di una grande ipocrisia, e tutto potete chiedermi meno che di essere un ipocrita. Per questo mi asterrò dalla votazione finale.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali